voglio essere preciso, ha preannunciato che chiederà al Consiglio dei ministri, credo riunito in queste ore, di esprimersi sulla volontà di porre la fiducia sul disegno di legge finanziaria.

potrà o dovrà vertere prevalentemente, se i senatori lo consentono, sulle questioni che riguardano il bilancio: Esaurita la discussione con questa accortezza, vi sarà la replica del relatore, senatore Tecce, e del Governo; poi passeremo all'esame degli articoli e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

nell'ambito del contingentamento previsto, ma con molta attenzione, una discussione ampia sul maxiemendamento che - credo

molti morti e feriti. Soprattutto, quel 12 dicembre ha rappresentato l'inizio della strategia della tensione, che ha colpito molto la nostra democrazia e ha lasciato una striscia di sangue.

colleghi senatori, il disegno di legge di bilancio n. 1184 al nostro esame è redatto a legislazione vigente. Il dibattito che si è svolto nella Commissione bilancio e le relazioni che abbiamo ricevuto dalle Commissioni hanno confermato in larga misura ciò che avevo affermato nella mia relazione in Commissione: il bilancio di previsione 2007, come modificato dalla manovra correttiva proposta dal Governo, corrisponde pienamente agli obiettivi programmatici contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria su cui ci siamo espressi a luglio e nella relativa nota di aggiornamento. Ciò risulta chiaramente anche dalla seconda nota di variazione di variazione trasmessa dalla Camera dei deputati, dalla quale risulta che il progetto di bilancio per il 2007 ha recepito sia le disposizioni del disegno di legge finanziaria come approvato dalla Camera dei deputati, sia le ulteriori norme introdotte con il decreto fiscale n. 262 del 2006, approvato in quest'Aula come collegato alla legge finanziaria. finanziaria. Nei primi articoli del provvedimento si definiscono lo stato di previsione dell'entrata (tabella 1) e poi lo stato di previsione del pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007. Si definisce poi l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a ripartire con propri decreti fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero stesso per l'anno 2007. Si definisce altresì l'importo massimo dei titoli pubblici da emettere in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in 55 milioni di euro. Si definiscono inoltre le cosiddette spese obbligatorie e d'ordine con apposito elenco. Ebbene, rispetto a ciò, rimandando al testo scritto per una serie di approfondimenti, vorrei sintetizzare che il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 evidenzia i seguenti importi di competenza, al netto delle regolazioni contabili e debitorie dei rimborsi IVA: le entrate fiscali si attestano a 431,4 a 431,4 miliardi, mentre le spese finali si attestano a 454 miliardi. Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali, risulta in termini di competenza, e al netto delle relazioni contabili e debitorie dei rimborsi IVA, pari a circa 23 miliardi di euro. La previsione del bilancio registra una forte riduzione del saldo netto da finanziare anche rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, derivante dall'aumento delle entrate finali. Anche il risparmio pubblico registra rispetto alle previsioni assestate per il 2006, che avevano un valore negativo, un miglioramento di circa 18 miliardi di euro, dovuto essenzialmente all'incremento delle entrate correnti per oltre 22 milioni di euro e alla riduzione di 3.240 milioni di euro delle spese correnti. L'avanzo primario, pertanto, registra un notevole incremento di 20.585 milioni. Questa tendenza all'aumento delle entrate sembra consolidarsi ancora nel 2007 anche se, ovviamente, non ha effetto su questa proposta di bilancio, per motivi evidenti legati alla legislazione vigente. È pur vero - e mi rivolgo anche ai colleghi dell'opposizione

anche per sollecitazione dell'opposizione immediatamente raccolta dal presidente Morando e dal Vice ministro. È un fatto certamente positivo, da non minimizzare ma da non enfatizzare, perché ovviamente vanno verificati i caratteri strutturali di tale aumento delle entrate fiscali, che pure ovviamente risponde ad una precisa strategia di lotta all'evasione. C'è ovviamente un dissenso, un diverso giudizio tra maggioranza e opposizione su come utilizzare queste entrate. È stato oggetto del dibattito in Commissione e sono certo lo sarà in Aula. Addirittura, secondo alcuni interventi, queste entrate avrebbero permesso permesso di ridurre gli aspetti strutturali, quantitativi e qualitativi, della manovra finanziaria stessa. Ovviamente non sono d'accordo. Tuttavia si tratta di un fatto nuovo ed importante perché risponde ad una precisa strategia del Governo. Da più parti - affronto un'altra questione - è stata sollecitata nel dibattito una rapida modifica degli strumenti, dei tempi e delle procedure di esame del bilancio e della legge finanziaria. Ovviamente nel dibattito non è emersa ancora una soluzione. Se ne parla ad ogni finanziaria. Mi limito, quindi, in qualità di relatore, a sottolineare che effettivamente è un tema che la stessa Commissione bilancio potrebbe, soprattutto se supportata dal parere dell'Aula, decidere di approfondire eventualmente in maniera congiunta con quella della Camera dei deputati, dato che il tema è stato richiamato in ogni intervento, sia in Commissione sia nel dibattito pubblico tra le forze politiche, soprattutto per quanto concerne l'abbreviamento dei tempi e la semplificazione della materia. Sostenere che sia stata già prospettata in Commissione una soluzione mi sembrerebbe eccessivo ed ottimistico, ma è assolutamente giusto sottolineare l'unanimità dell'esigenza di andare ad una riflessione e ad un cambiamento. Infatti, vorrei svolgere una breve riflessione: le regole che guidano la formazione e l'approvazione del bilancio riflettono sempre l'equilibrio di poteri che in un certo periodo storico ed in un determinato sistema istituzionale si realizza in materia di politica fiscale tra Parlamento e Governo. Nel nostro sistema istituzionale l'articolo 81 della Costituzione attribuisce al Parlamento il potere di approvare il bilancio dello Stato, pur riservandone la presentazione al Governo. Dal punto di vista dell'entrata, l'articolo 23 della Costituzione prevede che qualsiasi prestazione personale o patrimoniale possa essere imposta solo per legge. Dal lato della spesa, l'azione del Parlamento sul bilancio indica la priorità dell'azione pubblica e diventa un limite alla discrezionalità dell'Esecutivo nella gestione delle risorse. In tale contesto, il principio di specificazione, cioè la definizione dell'unità di voto parlamentare, diventa l'elemento da prendere in considerazione per comprendere come il Parlamento, di fatto, vincoli l'azione del Governo. Infatti, la legge n. 94 del 1997 e il decreto legislativo attuazione n. 279 del 1999, prevedevano interventi riformatori in materia che hanno determinato un riordino dei capitoli di bilancio, individuando, come ben sanno i senatori, nelle unità previsionali di base Le u.p.b. costituiscono aggregazioni di risorse finanziarie, attribuite ad un centro di responsabilità amministrativa, ossia la responsabilità di un dirigente. La presentazione della spesa per centri di responsabilità viene accompagnata da una classificazione per funzioni-obiettivo. Nell'attuale decreto legislativo si passò da 6.000 capitoli a circa 1.500 u.p.b. del bilancio attuale. Si è trattato quindi di una riorganizzazione che, da un lato, ha ridotto in modo significativo il livello di dettaglio della decisione parlamentare, dall'altro ha introdotto la distinzione tra bilancio politico e bilancio gestionale, tra funzione di indirizzo e di controllo dell'organo politico e funzione di gestione affidata ad una struttura dirigenziale. Rimando al testo scritto per alcune riflessioni più articolate in questa materia. Voglio soltanto dire che l'esperienza degli anni più recenti ha visto emergere, a mio avviso in maniera preoccupante, un binomio «flessibilità-riduzioni di spesa». La concessione ai Ministeri di spesa di una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse ha costituito nei fatti la contropartita alle iniziative di contenimento della spesa, che continua anche in questa finanziaria. Con l'articolo 22, comma 21, del disegno di legge di bilancio che stiamo esaminando, sono rese possibili compensazioni di cassa, nell'ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle u.p.b. del medesimo stato di previsione. A tal proposito voglio informare l'Aula che come relatore ho proposto un emendamento, approvato dalla Commissione, che obbliga il Governo ad informare le competenti Commissioni parlamentari dei decreti di variazione compensativi nell'ambito di ciascun titolo di bilancio tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione. previsione. Rimandando, ripeto, al testo scritto, vorrei arrivare ad alcune conclusioni. In primo luogo, ritengo sia molto importante, in linea con l'obiettivo di una migliore trasparenza della decisione di bilancio, intervenire sul disegno istituzionale delle strutture che forniscono il supporto tecnico alle decisioni di politica fiscale. Negli ultimi anni è più volte emersa l'esigenza di fare il punto sulla gestione in corso di esercizio si è parlato di ciò anche in Commissione - attraverso un sistema di monitoraggio e un affidabile aggiornamento delle previsioni. Personalmente desidero sottolineare la novità rappresentata dall'introduzione di uno schema di «bilancio ambientale» all'interno del disegno di legge di bilancio. In proposito mi permetto di avanzare una riflessione: vanno enormemente valorizzati tutti gli strumenti che permettono una lettura sintetica del bilancio ed una sua semplificazione. Tali strumenti sono utili sia per il controllo che per l'indirizzo del Parlamento, sia per la possibilità di comunicazione con i cittadini. Ovviamente mi riferisco a tutta l'elaborazione relativa al tema del bilancio sociale, inteso non soltanto come bilancio per gli effetti contabili ma anche per gli effetti sociali che determina, sapendo che il bilancio sociale, che analizza le spese per obiettivi aggregati e risultati visibili, è la premessa del dibattito aperto sul bilancio partecipativo.

Ritengo che questo bilancio, che abbiamo discusso e approvato in Commissione, sia funzionale a una finanziaria che afferma l'obiettivo strategico di una contestualità tra interventi di risanamento, equità e sviluppo, mantenendo pienamente l'impegno mantenendo pienamente l'impegno assunto in sede europea di un rapporto tra indebitamento e PIL sotto il 3 per cento visti i dati, anche sotto il 2,8 per cento stimato all'inizio della manovra - grazie all'inizio di ripresa strutturale e all'aumento delle entrate fiscali su cui mi sono soffermato. Si ricostituisce finalmente un avanzo primario che non c'era più; ora bisognerà puntare di più sulla crescita e lo sviluppo partendo da chi lavora, permettendo l'espansione della base produttiva, unico modo per rilanciare anche la domanda interna e l'esigenza dei più deboli, dei più poveri, degli incapienti, la cui esigenza di inclusione sociale in questa finanziaria, per unanime giudizio, non trova ancora un adeguato spazio, e per affrontare un problema di civiltà e di affermazione di quei diritti di cittadinanza, che sono anche una condizione di sviluppo economico equilibrato e socialmente sostenibile. Il bilancio, insomma, fotografa e permette di dire che su questa linea si può andare avanti; dipende dal Parlamento, dipende dal Senato

È noto che la 5a Commissione, lo ha detto il presidente Marini, non ha concluso l'esame della finanziaria, vorrei però pubblicamente ringraziare il presidente Morando per il grande lavoro fatto, per l'equilibrio, riconosciuto anche dall'opposizione, con cui ha guidato il nostro lavoro e la serietà che ci ha condotto ad approfondire molti temi e a fare un dibattito di cui sono certo il Governo vorrà tener conto. Ci sono testi, dibattiti e proposte, da questi bisogna partire. Insieme al Presidente, vorrei ringraziare tutti i colleghi della Commissione bilancio, di opposizione e di maggioranza. Vorrei ringraziare il senatore Morgando, che ha svolto il suo ruolo di relatore della finanziaria, gli uffici della Commissione e tutti gli uffici del Senato, che ci hanno per quindici giorni supportato e sopportato. Non spetta a me dire ciò che si farà e ciò che sarà deciso dal Governo e dal Parlamento; quel che vorrei dire è che il lavoro fatto è patrimonio del Senato e da qui si deve partire per provare a bilanciare le esigenze di una finanziaria rigorosa con le esigenze di crescita dei cittadini e di tutta la nostra società.

non ha concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria nei tempi che lei, signor Presidente, ci aveva assegnato. Per queste ragioni, questa mattina il relatore Morgando non terrà la relazione di maggioranza,

(e, soprattutto, anche se l'avessi, non avrei il potere) di sostituirmi a lui nel fornire all'Aula valutazioni politiche sui contenuti del

Dicevo che non ho alcuna intenzione, né il potere di sostituirmi al senatore Morgando nel fornire all'Aula valutazioni politiche sui contenuti della legge finanziaria.

di legge finanziaria. Anche la Commissione bilancio del Senato, in seconda lettura, non ha concluso i suoi lavori. Da ciò deriva, colleghi, una conseguenza

la legge finanziaria 2007 sarà approvata senza un compiuto esame tecnico-politico in Commissione. cosa s'intende per «compiuto esame»? Vuol dire un esame compiuto a partire dalle diverse opzioni politiche che la maggioranza e l'opposizione, in tema di politica economica, presentano al Paese, ma significa anche un esame compiuto sotto il profilo tecnico, della tecnica finanziaria e della tecnica giuridica;

600 persone. Da questo punto di vista, non c'è dubbio che ci troviamo in presenza del rischio assai serio serio che l'esame tecnico delle norme, che traducono in legislazione le volontà politiche, le scelte alternative di politica economica, sia tale da inficiarle, in una certa misura, per mancanza di fondamento giuridico, di correttezza tecnica. Dopo un compiuto, attentissimo esame in Commissione, la mia opinione personale è che in Aula, fatte salve le

quella del Ministro del tesoro britannico che, in un certo giorno di settembre, scende a Westminster con una valigetta in mano, dentro la quale c'è il progetto di *budget*

perfetto meccanismo di decisione di bilancio che ammiriamo in tutto il mondo. Cosa succede nei trenta giorni precedenti?

si sviluppa un confronto intenso, secondo lo schema classico della democrazia inglese di dura contrapposizione tra maggioranza e opposizione, sulle proposte alternative. Terminato questo lavoro che dura un mese, il Governo - come si usa dire - fa sue le carte, prende atto del lavoro parlamentare, che non ha modificato il progetto, ma ha proposto di modificare il progetto, torna a riunirsi, approva un disegno definivo di *budget* e, a quel punto, ecco l'immagine del Ministro che arriva con la valigetta a Westminster e dopo cinque giorni ne esce con il *budget* approvato. Ora, badate che la cosa è semplicissima: se vogliamo affrontare veramente il tema della sessione di bilancio e della sua riforma, dobbiamo guardare, prima di tutto, al lavoro delle Commissioni e, in particolare, a quello delle Commissioni bilancio. Poi, in una certa misura, in Aula è inutile strapparsi continuamente le vesti:

violazione di non so quale regola democratica perché si era scelto di mettere la fiducia; adesso, le parti sono cambiate, ma i lai sono gli stessi, gli argomenti sono identici e così via. Il problema, però, secondo me (lo dico molto modestamente, ma lo faccio perché ne sono profondamente convinto), non è che a un certo punto, svolto il lavoro di approfondimento tecnico-politico nelle Commissioni, l'Aula (della Camera o del Senato) sia chiamata a votare sì o no - prendere o lasciare - sui risultati di questo lavoro:

votare sì o no su un disegno di legge compiuto, misurato, valutato in ogni suo singolo aspetto, alla fine di un processo di decisione, in un certo senso, è normale; anzi, ritengo che sia più democratico che impegnare 600 persone in centinaia e centinaia di votazioni su singole proposte di modifica.

è in Commissione, però, che si devono conchiudere l'approfondimento e la valutazione tecnica, oltre che politica. Allora,

è la seguente: se vogliamo uscire dall'*impasse* in cui ci stiamo progressivamente cacciando, a mio avviso, con un'esagerata e irresponsabile *nonchalance*, da parte di opposizione e maggioranza (e la cosa non è di oggi, ma viene da lontano), credo che dobbiamo lavorare immediatamente a un mutamento delle regole della sessione di bilancio, affinché questa abbia al suo centro i lavori delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

una relazione, funzionale ad una discussione tra maggioranza e opposizione, sulle regole della sessione di bilancio (l'oggetto è il combinarsi della legge di contabilità con il Regolamento del Senato), Senato), tale da consentire, alla fine di quello stesso mese, ai diversi Gruppi, ai diversi parlamentari e, naturalmente, anche al Governo - se lo riterrà - di presentare disegni di legge di modifica della legge di contabilità

Alla fine di gennaio, se questi disegni di legge e proposte saranno stati formulati, si potrà poi, nel mese immediatamente successivo, provare a definire una soluzione. La seconda indicazione di lavoro che viene, signor Presidente, per noi è una conferma, perché ne abbiamo già parlato in occasione della discussione sul bilancio del Senato. La centralità del Parlamento, che io in quanto governista da sempre credo che sulla decisione di bilancio vada confermata,

autonomia tecnica, una forte autonomia rispetto alla capacità di analisi e di valutazione tecnica che ha il Governo sulle scelte finanziarie

viene davvero valutato nei suoi effetti finanziari solo dalla Ragioneria generale dello Stato, perché solo essa ha le competenze tecniche necessarie per poterlo fare. O noi abbiamo un ufficio del bilancio del Parlamento che abbia la stessa autorevolezza, la stessa affidabilità, la stessa dotazione di capacità tecniche che hanno gli uffici del Governo o non ne verremo mai a capo.

i principali giornali hanno dibattuto, come se si trattasse di una cosa tecnicamente possibile, del fatto che si starebbe discutendo di usare delle risorse di parte capitale

è possibile che per poter affermare questa elementare verità bisogna che parli il ragioniere generale dello Stato perché il Parlamento a casa

la capacità di autorevolmente garantire che cose di questo tipo non sono nemmeno proponibili (e, infatti, non sono state proposte, intendiamoci bene). È un piccolo segnale di un fatto generale. L'autonomia

non hanno la quantità, la solidità, non hanno la capacità di coordinamento necessaria. Allora bisogna passare subito,

consenta di soffermarmi anche sull'intervento del presidente Morando in ordine alle determinazioni che il Senato può assumere per una più efficace sessione parlamentare di bilancio. In Commissione l'opposizione ha lavorato altrettanto seriamente, e gli atti possono facilmente evidenziare quanto sia stato forte l'impegno su alcuni temi di grande rilievo.

Anzi, esso fornisce il pretesto, in senso positivo, per una revisione della sessione di bilancio che la Commissione

per poter dire al Paese che il Parlamento si concentra sui grandi temi e occupa il 95 per cento del suo tempo in Commissione per affrontarli, emendarli e discuterli.

la definizione di strumenti che consentano un'efficace discussione nelle Commissioni e un grande dibattito politico sulle alternative di politica economica e finanziaria in Aula sia un obiettivo da discutere e auspicabilmente conseguire. Mi sembrava utile che l'opposizione fornisse queste poche note di commento alla relazione del presidente Morando per assicurare che prendiamo in seria considerazione

Come è noto, presidente Marini - mi rivolgo a lei perché è il nostro supremo difensore - il Governo ha presentato in Commissione bilancio una tabella palesemente sbagliata. Sbagliata, signor Presidente, non per cifre di modica entità (consentitemi questo passaggio con qualche allusione). Noi già siamo contrari alle modiche entità,

nella migliore o nella peggiore delle ipotesi, dimenticava di inserire dinanzi alla Commissione bilancio un'entrata di 8 miliardi di euro.

Abbiamo preso atto del ravvedimento operoso del vice ministro Visco ed abbiamo preso atto che il ministro Padoa-Schioppa, perlomeno dinanzi al Parlamento, non se n'era accorto,

Detto questo, signor Presidente, dato che nella tabella si era passati dal 16 novembre al 30 novembre, le nuove entrate in più erano di nuovo di ulteriori 4 miliardi. In altri termini, è bastato il trascorrere dal 16 al 30 novembre per un ulteriore aumento di 4 miliardi.

di affermare sottovoce (noi, però, lo abbiamo ascoltato lo stesso) che con l'autotassazione aumenterà ancora il *surplus* di tasse. Signor Presidente, non è inverosimile

il settimo anno da quando un malore ha sottratto a questo Parlamento e al dibattito nel Paese una delle menti più brillanti e più oneste della Prima e della Seconda Repubblica;

vicino a quest'Aula, ha sollevato, in un ragionamento pubblico collettivo, la necessità di introdurre nel Parlamento italiano un meccanismo simile al *Congressional budget office* americano, cioè uno strumento tecnico indipendente per consentire al Parlamento, ai deputati e ai senatori,

che fa assumere una responsabilità istituzionalmente non corretta nelle mani esclusive dell'Esecutivo che, con maxiemendamenti e fiducia, chiede il voto ai parlamentari senza che questi, sia della maggioranza sia dell'opposizione, abbiano la possibilità di capire con esattezza e correttezza ciò che andranno a votare, a favore o contro.

non sono state compiute, ma non è del tutto vero che non siano state fatte. Le conclusioni alle quali siamo giunti ieri, che non completano il lavoro in modo tale da poter riferire in modo corretto ed istituzionale in Aula, non possono farci dimenticare quanto è emerso sul piano tecnico e sul piano politico ed è bene che di ciò l'Aula venga compiutamente informata. Cosa è emerso sul piano tecnico che giustifica la richiesta del presidente Morando di attrezzare gli uffici come organo indipendente a supporto del Parlamento?

Ricordo solo, per brevità di tempo, che abbiamo aperto la legislatura con la questione dell'IVA sugli immobili

perché non conteneva la stima di 13 miliardi di gettito che sarebbero stati conseguenti a quel decreto. Il Governo, giustamente, disse che gli uffici si erano sbagliati e corresse il decreto nel momento della conversione.

chiedemmo in Commissione la disponibilità dei dati sulle entrate delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2006. Quei dati sono fondamentali per poter proporre all'Aula il bilancio di previsione per l'anno 2007. Il Governo ha presentato una prima tavola, risultata sbagliata, e, ieri mattina, ne ha presentata una seconda dalla quale dalla quale emerge che il bilancio che è stato presentato a quest'Aula contiene numeri falsi, non veri, non per ammissione di qualche esperto o di qualche componente dell'opposizione, ma per ammissione del Governo è un fatto che non è mai avvenuto nella storia della Repubblica italiana. Il Governo ieri ha detto che i dati delle entrate delle pubbliche amministrazioni per il 2006 arriveranno a fine anno

numeri, afferma che dei 34 miliardi al 30 novembre soltanto 8 possono essere considerati delle *una* *tantum* non riproducibili nelle tabelle per l'anno 2007. almeno 25 miliardi: l'aumento del gettito IRPEF dei lavoratori dipendenti e autonomi, l'aumento del gettito dei contributi sociali, l'aumento del gettito IVA, tutti incrementi di gettito legati alla ripresa dell'economia e all'emersione del sommerso che hanno portato ad un *boom* di occupazione, magari flessibile, ma regolare, che paga IRPEF e contributi. Il Governo ha che nel 2006 è avvenuto un fatto importante: 25 miliardi di quel maggiore gettito sono strutturali e permanenti, a meno che non ci sia un retropensiero e cioè, come noi sosteniamo, che l'attuale finanziaria ucciderà la ripresa economica, abbatterà la crescita economica e allora quelle entrate non ci saranno proprio per colpa della finanziaria. Ma se così non è, come auspicheremmo, la tabella delle entrate del bilancio che ci apprestiamo a discutere e a votare, signor Presidente, contiene un numero falso per ammissione

masochismo e sadismo con il quale viene poi a proporre una legge finanziaria che incrementa ulteriormente le tasse, quindi le entrate delle pubbliche amministrazioni, di altri 35 miliardi a valere sul 2007. Ma la ragione politica

perché esso non risponde né alle esigenze del Paese, né alle disposizioni contenute nella legge di contabilità. Si tratta di un dibattito un po' sterile, che ogni volta appassiona pochi di noi, ma che ha un'enorme importanza perché il bilancio dello Stato

possa disporre ed inviare alla Corte dei conti per la registrazione le variazioni compensative in termini di cassa. Presidente, non si possono fare compensazioni con una disposizione all'interno del bilancio tra diverse unità previsionali di base: ciò è assolutamente contrario alla legge di contabilità. Non solo, ma non si può dare un'autorizzazione ad operare le variazioni senza

21 dell'articolo 22 del disegno di legge di bilancio è ripetuto nella legge finanziaria al famoso e famigerato, per la discussione che abbiamo svolto in Commissione, comma 53 dell'articolo 18.

vengono definiti i criteri e le modalità per le riduzioni e i trasferimenti». Quindi, a questo punto, se lo si stabilisce con la legge finanziaria che è la sede opportuna per poterlo fare, non lo si può fare con la legge di bilancio, e pertanto l'attuale legge di bilancio è contraria alla legge di contabilità.

disposto come prerogativa al Governo nella legge di bilancio debba essere inviato all'esame del Parlamento e delle competenti Commissioni parlamentari. Ma le Commissioni parlamentari effettuano una vigilanza

è da lungo e da troppo tempo nel Paese e in Parlamento - trova la principale responsabilità oggi nella maggioranza e nel Governo. Infatti, signor Presidente,

visto che in una giornata lavorativa di 12 ore esistono 720 minuti, si possono esaminare 1.000 emendamenti e quindi in cinque giorni, 5.000 emendamenti. Lei mi dirà «ma perché presentare 5.000 emendamenti?». Va bene, allora discutiamo 1.000 articoli. Ma si può togliere al Parlamento la necessità e il diritto di discutere per cinque minuti di ogni articolo della finanziaria? E c'è bisogno sempre di sette o otto giorni, non è il tempo disponibile che il Governo ha concesso con una finanziaria vastissima, enorme che vuole presuntuosamente affrontare tutti i problemi del Paese, senza risolverli. Ma c'è di più. Il Governo, venendo in Commissione, non ha accettato una discussione. E la maggioranza, signor Presidente - è bene che il Parlamento ed il Paese lo sappiano - ad un dato momento doveva continuamente sospendere la seduta, sino a quando si è realizzato, con il minimo di esperienza che i commissari hanno per i lavori della Commissione, quello che ha denotato il fallimento dei lavori dei lavori parlamentari già da venerdì: siamo rimasti attoniti come i giapponesi, in quanto non sapevamo che la finanziaria non si poteva completare in Commissione. Abbiamo continuato a fare una guerra,

la Costituzione materiale e il Parlamento, invece di rappresentare la centralità della democrazia nel Paese, ha finito per non rappresentarla più. E quando la maggioranza

che sabato e domenica, quando hanno capito che gli emendamenti consegnati ai componenti della maggioranza non avevano la possibilità di essere discussi, hanno cominciato a venire in Commissione anche senza cravatta,

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, questa mattina

concludendo amaramente che la stessa Commissione non ha potuto concludere l'esame del bilancio che ci è pervenuto dalla Camera. Non ha potuto cioè compiere quell'esame tecnico e politico che garantisce non soltanto la dialettica democratica tra maggioranza e opposizione, ma nemmeno quella ricognizione di carattere tecnico che consente di migliorare normativamente e legislativamente il testo. Perché è successo questo? Si potrebbe dire da questa parte, anche con enfasi, che sono stati presentati

per complessivi 177 emendamenti determinanti perché provenienti dal Governo e dal relatore di maggioranza, quindi incisivi, in grado cioè di modificare sostanzialmente la finanziaria.

Governo. Se ci si sofferma sui 2.000 emendamenti del centro-sinistra e su quelli successivi del Governo e del relatore, oltre a tutto il dibattito che si è svolto alla Camera, ben si comprende come la finanziaria

Ce la potremmo cavare con questi dati e dire che se non si è arrivati a definire un testo e se non si è arrivati a far compiere al Parlamento quell'esercizio delle sue competenze questo si deve agli errori, all'auto-ostruzionismo o in qualche modo alla farraginosità delle norme che il Governo ha varato con la finanziaria. A questa

conseguentemente, a quanto è stato detto, ed ulteriormente modificato l'andamento dei lavori. Ma non è questo che mi preme rilevare in tale fase; tale fase; sarebbe una liturgia stanca, una liturgia del gioco delle parti che comunque non risolverebbe il il grave problema che abbiamo di fronte e che questa mattina ha riguardato proprio l'intervento del Presidente della 5a Commissione. È vero, è stato sconfitto il Parlamento. Ha detto bene non un membro dell'opposizione, non lo dico io, ma il Presidente della 5a Commissione che è stato sconfitto il Parlamento. Chi ha coscienza democratica non può non riconoscere che quando uno dei provvedimenti legislativi più importanti di un'attività legislativa che si compie in un anno non raggiunge il suo completamento, siccome esso incide profondamente sugli equilibri economici e sulla situazione sociale del Paese incide profondamente sullo sviluppo del Paese, ben si comprende come il ruolo del Parlamento diventi secondario, subordinato al ruolo dell'Esecutivo. La nostra Costituzione prefigura una Repubblica parlamentare, un primato del Parlamento sull'Esecutivo. In questi termini, invece, si rovesciano i valori costituzionali, perché il primato diventa del Governo e lo diventa ancor più nel momento in cui poi pone anche in questa Aula una fiducia alla quale accederà un consenso militarizzato della maggioranza.

Certo, si è detto da più parti: «Modifichiamo la legge di contabilità finanziaria». Certamente le regole possono aiutare, ma qui vi è una questione politica. In passato, anche con un numero maggiore di emendamenti, si è potuto svolgere e completare il lavoro della 5a Commissione e il Parlamento ha potuto esercitare la sua funzione, perché c'era un di più di politica. Oggi nel Paese c'è un dibattito esterno al Parlamento, sicuramente esterno alla Commissione bilancio, che ha una portata così forte di contrapposizione e di scontro ideologico che condiziona enormemente un sereno e costruttivo dibattito tra maggioranza e opposizione. Di chi la responsabilità di questo clima di scontro che c'è nel Paese? Ciascuno si metta una mano sulla coscienza; ognuno ha una sua parte di responsabilità; sta alla politica più avvertita, a quella con una sensibilità che riguardano la democrazia del Paese, ma anche ai contenuti di carattere economico e sociale che sottostanno ai grandi temi della democrazia,trovare

dell'efficienza del nostro sistema politico e di come si possa trovare una via d'uscita. Egli ha posto un interrogativo al Paese e alle coscienze più sensibili sui temi della democrazia. Non si può lasciar

situazione a legislazione vigente, non fa che riportare le partite attive e passive esistenti. Vi sono invece - lo abbiamo indicato in modo specifico

sufficiente attenzione - la relazione e il grido di dolore del Presidente della Commissione bilancio. Sulle questioni che riguardano il *de* *iure* *condendo*

hanno un presupposto indefettibile: che esista cioè un Governo omogeneo, non dico nel quale tutti la pensino allo stesso modo, ma dove comunque vi sia una base comune di lavoro e di valori e una maggioranza omogenea.

un peso e un'incertezza considerevoli, con una moltiplicazione di articoli, o meglio di commi, ognuno dei quali dovrebbe rappresentare un articolo, come mai si era visto nella nostra legislazione. A questo proposito, Presidente, vorrei ricordare una sollecitazione che l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - che è qui presente

esame: «Con l'occasione, ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta» udite udite - «di 49 commi» (oggi parliamo di 810 commi) «e occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria» - cioè il messaggio di rinvio alle Camere - «per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare, invalso da tempo, che non appare coerente con la *ratio* delle norme costituzionali che disciplinano il procedimentolegislativo e, segnatamente, con l'articolo 72della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e convotazione finale».

in questa e in analoghe materie, come la decretazione d'urgenza, dove si pensava che tutto rientrasse negli *interna corporis* e che fosse precluso l'intervento della Corte costituzionale, tanto si tirò la corda e si arrivò a usare gli strumenti legislativi in maniera impropria, che alla fine la Corte costituzionale dovette intervenire. Oggi siamo di fronte a un disegno di legge, Presidente, che contiene, oltre ai primi 17 articoli in parte corposi, un diciottesimo articolo composto di 810 commi, fatto mai avvenuto nella storia del nostro Parlamento. Abbiamo assistito - lo riconosco - a una degenerazione nella presentazione di testi legislativi, ma in questa materia, come in altre, la quantità diventa qualità, quando si eccedono certi limiti. Dobbiamo aspettarci che il maxiemendamento che il Governo presenterà

che vada fatta una riflessione approfondita, perché la certezza del diritto, che viene meno con questo tipo di legislazione, è un valore precondizione di qualsiasi Stato liberaldemocratico: non può esistere uno Stato liberaldemocratico se non è anche uno Stato di diritto, cioè fondato sulla certezza delle norme giuridiche, ma ancor prima

Ancor prima, Presidente - e qui richiamo la sua sensibilità e responsabilità istituzionale - è questo Parlamento, nel momento genetico della legge, che non è in grado di conoscere

ha superato ogni limite. Ma perché si è arrivati a tali conclusioni? Perché la finanziaria è diventata il veicolo di tutto e del contrario di tutto,

non si è potuto esaminare in Commissione per i noti motivi di sospensione dei lavori.

Illustrerò, signor Presidente, argomenti che ella ha avuto la pazienza di ascoltare in uno scambio informale che io mi sono arrogato (forse con troppo arbitrio) di instaurare con lei. Non farò riferimento a quei documenti perché conosco le regole, signor Presidente, tuttavia la validità del contenuto degli stessi rimane tanto nella mia, quanto nella sua memoria. Con senso

cominciando a dirle e a dire all'Aula che riteniamo che il disegno di legge finanziaria 2007, con prevalente e specifico riferimento all'articolo 18, commi 206 e 207, sia inficiato da gravi profili di contrasto rispetto a precetti normativi e a regolamenti vigenti. Il quadro di confliggenza di cui trattasi può essere così compendiato: confliggenza rispetto ai dettati della Costituzione, in particolare definiti dagli articoli 70 e 76 della suprema Carta; confliggenza rispetto alla legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato; confliggenza rispetto al Regolamento del Senato che esclude la possibilità, signor Presidente, che tale Aula parlamentare venga o possa essere interessata da proposizioni e/o domande del Governo dal contenuto e dalla forma improponibili. ora ad illustrare i tre motivi di confliggenza. Quanto alla confliggenza rispetto ai dettati della Costituzione, è dato convenire, da chiunque si faccia guidare da coscienza autonoma, libera, serena, responsabile, verso il bene comune, che il combinato disposto degli articoli 70 e 76 della norma costituzionale non consente di dedurre, o anche soltanto di far balenare la possibilità, che il diritto al bilancio sia prerogativa non esclusiva del Parlamento, ma anche concorrente del Governo, una concorrenza realizzabile, magari, mediante l'istituto della delega.

La delega al Governo, dunque, realizza il contenuto dei commi 206 e 207 dell'articolo 18 del testo della finanziaria. delega piena, posto che delle indicate quote accantonate per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, al comma 206 in discorso, nonché degli ulteriori accantonamenti di cui al successivo comma, nulla più saprà (o saprebbe) il Senato, giacché la destinazione e la gestione di tali accantonamenti è demandata al Ministro dell'economia e delle finanze che le porrebbe in essere a mezzo di suoi decreti. Una delega piena, cui corrisponderebbe, ove venisse assentita e resa possibile da un'ostinata scelta politica, un crimine ai danni del principio della Carta costituzionale, che vuole, ripeto, con l'articolo 76, che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo». Quanto al secondo motivo di confliggenza, quello rispetto alla legislazione vigente, pare del tutto palese che le disposizioni oggetto dei presenti rilievi contrastino con talune strutture portanti della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni Talune di tali strutture possono essere indicate come segue, volendo seguire un criterio di estrema sintesi. La finanziaria provvede per il periodo annuale considerato «alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente

Pertanto la norma, vista in un quadro di interrelazione e di sistematicità con altre disposizioni contenute nella medesima legge n. 468 del 1978, enuncia la necessità che le indicate quote annuali accantonate vengano esposte al Parlamento sia nella loro formazione, sia nella loro specifica e articolata utilizzazione, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009. Tocca constatare e denunciare che nella formulazione della disposizione della finanziaria non vi è traccia né dell'una, né dell'altra specificazione

che descrive l'accertamento fatto dal Presidente dell'Assemblea, sentita la 5a Commissione permanente, non può essere avulso, signor Presidente, signor Presidente, da una considerazione di buon senso e di comune ragionevolezza. Al Senato e ai singoli parlamentari non possono e non debbono essere sottoposti atti e documenti dai contenuti improponibili per manifesta incostituzionalità e per palese e multipla illiceità, che contrastano con le norme che regolano la contabilità di Stato, come nel caso dei citati commi 206 e 207 dell'articolo 18 per i quali sarebbe stato opportuno, a nostro avviso, proporre lo stralcio già prima dell'assegnazione del testo alla Commissione di merito. Poiché ciò non si è verificato e senza voler entrare nel merito delle responsabilità o delle omissioni, tocca far constare, per per l'intanto, che il Senato è esposto al rischio di varare un testo legislativo privo di contenuto e di natura a valenza effettivamente legislativi. Vale a dire, il Senato viene impegnato in un'attività offensiva Un'altra occasione mancata di buon servigio al bene delle istituzioni democratiche e della stessa democrazia. Un'occasione di ulteriore e mancato discernimento fra ciò che è bene e corretto, da ciò che bene e corretto non è. Un'altra Un'altra prova di distrazione o fors'anche di stoltezza nel non aver colto che si può e si deve essere tutti concorrenti, ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie posizioni politiche, nel rispettare le regole. Così, per essere concorrenti della tenuta della democrazia e del suo consolidamento su piani sempre più alti, diversamente, non resta

che non può esser normato attraverso la legge finanziaria e che merita certamente di essere aggiornato e magari riformato attraverso il dibattito parlamentare e il lavoro di Commissione, con una legge ordinaria

premesso, la disciplina relativa all'obbligo scolastico trova fondamento nel precetto dell'articolo 34 della Costituzione, che garantisce per almeno otto anni l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore, senza porre limiti temporali al suo svolgimento. In base al dettato costituzionale deve ritenersi garantito un certo percorso d'istruzione, individuato in termini temporali, ma non può invece considerarsi garantito il risultato scolastico, sì che appaiono generalmente e pienamente legittime le disposizioni relative all'adempimento dell'obbligo scolastico e al proscioglimento da esso, a condizione che siano emanate con norme di rango primario. Le norme contenute negli articoli 110 e 112 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano l'istruzione inferiore con disposizioni comuni alla scuola elementare e media (attualmente denominate scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) individuano nei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età coloro che sono soggetti all'obbligo scolastico. Il sistema delineato nelle predette norme configura l'istruzione inferiore anche come un dovere che deve essere assolto nel citato periodo d'età, e dal quale si è prosciolti se al compimento del quindicesimo anno d'età non sia stato conseguito il diploma di licenza media, ma siano state osservate per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico. Trascorso il periodo durante il quale è obbligatoria la frequenza scolastica, l'istruzione inferiore perde l'originaria configurazione di dovere e il relativo diritto può essere esercitato mediante la frequenza di corsi per adulti, finalizzati al conseguimento della licenza elementare e della licenza media, come previsto dagli articoli 137 e 169 dello stesso decreto legislativo n. 297 del 1994. Il diritto-dovere introdotto dal modello della Moratti ha modificato gli assetti ordinamentali attraverso la tipologia dei percorsi scolastici formativi, rispondendo puntualmente agli appelli dell'Europa di prolungare l'obbligo d'istruzione, attraverso l'inserimento della VET (*Vocational Educational Training*). La legge n. 53 del 2003, la cosiddetta legge Moratti, ridefinisce ed amplia con decreto legislativo n. 76 del 2005 l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'attuazione del diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni, ai fini del conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno d'età, si realizza a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione e mediante regolamenti adottati di concerto con la Conferenza unificata Stato-Regioni, prevedendo tra gli interventi del Piano programmatico interventi di orientamento contro la dispersione scolastica. Il predetto decreto legislativo n. 76 del 2005 è stato prorogato dal Ministro Fioroni di ulteriori 18 mesi riguardo ai termini per l'eventuale modifica. Orbene, la Legge Finanziaria, al comma 278 ridefinisce l'obbligo scolastico e innalza l'età minima per l'accesso al lavoro, disponendo che a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 l'istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine viene elevata a 16 anni l'età per l'accesso al lavoro. Il comma 279, autorizza, fino alla messa a regime della nuova disciplina, la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. Il Governo introduce nella Legge Finanziaria (che non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio), una disposizione che modifica l'obbligo scolastico, senza prima abrogare o comunque introdurre norme di raccordo con il decreto legislativo n. Si mantengono difatti in vita "i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale" previsti dalla Legge Moratti di intesa con le Regioni, prevedendo che strutture formative concorrano a svolgere percorsi e progetti idonei all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Detto contesto normativo e ordinamentale desta forti perplessità! La svolta federalista e, quindi, l'evoluzione costituzionale e legislativa assegna, poi, alle Regioni ampi poteri normativi, in materia d'istruzione e formazione professionale, definendo un'area di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. L'estensione dell'obbligo d'istruzione al primo biennio della scuola secondaria pone dei problemi in ordine alla compatibilità di tale provvedimento legislativo statale, peraltro privo di legittimità, con l'autonomia regionale in tema di Istruzione e Formazione Professionale. L'articolo 34 della Costituzione riguarda l'istruzione "di base". L'estensione dell'obbligo scolastico mediante ricorso all'obbligo formativo, fa *de facto* leva sul dovere sociale dello svolgimento di un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. L'articolo 4 si riferisce invece "al dovere di lavorare", e l'istruzione, anche quando si svolge nell'ambito di istituzioni della IeFP, non può essere considerata espressione di tale dovere. L'estensione dell'obbligo scolastico al di là dell'istruzione inferiore è incostituzionale, salvo che il legislatore non qualifichi anche il biennio delle attuali scuole superiori come facente parte dell'istruzione inferiore".

La scuola media o scuola secondaria di primo grado italiana, nell'ambito dei sistemi europei rappresenta l'unico ciclo medio che duri tre anni, dagli 11 ai 14 anni di età dell'alunno. In quasi tutti gli altri paesi la scuola media o secondaria di primo grado, sotto nomi diversi (college, educaciòn secundaria obbligatoria, comprehensive school, secondary school, gymnasios) o addirittura, come nei paesi scandinavi, sotto la forma di ciclo superiore della primaria o della scuola di base, dura quattro e/o copre un'età che va o dai 10 ai 15 anni (Germania), o dai 12 ai 16 (Spagna, Belgio, Scozia) o dagli 11 ai 16 (Inghilterra e Galles) o dagli 11 ai 15 (Francia, Svizzera) o dai 13 ai 16 (Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia) o dai 12 ai 15 (Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo). In un caso o nell'altro o coincide con la conclusione dell'obbligo scolastico a 15 o a 16 anni o si avvicina comunque di molto al 16° anno di età. Il superamento dell'arco temporale, indicato dall'articolo 34 della nostra Costituzione, ai fini dell'adeguamento ai citati Paesi dovrebbe essere effettivamente collegato all'acquisizione di competenze di base nell'arco del proprio percorso educativo. In secondo luogo, la scelta statale di delimitare la durata e la tipologia dell'istruzione obbligatoria inferiore, è vincolata al principio di leale collaborazione con le Regioni. Lo Stato non può ridefinire dal punto di vista temporale e contenutistico l'obbligo d'istruzione, senza tenere conto che la competenza legislativa in materia d'istruzione spetta alle Regioni, né che dell'istruzione, per volontà espressa dalla Costituzione fa adesso parte anche il sottosistema delle IeFP ( istruzione e formazione professionale). Le modalità scelte in merito alla questione dell'obbligo scolastico, impongono per lo meno la richiesta del parere obbligatorio della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge n. 400 del 1988 e dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. La formalizzazione di un'intesa con le Regioni si renderebbe, poi, necessaria, qualora la ridefinizione dell'obbligo di istruzione determinasse una contrazione delle attuali competenze regionali, in tema di istruzione e di IeFP. Ribadendo quindi le riserve circa l'incertezza legislativa,

che il TFR è un risparmio del lavoratore che nel passato veniva messo nelle disponibilità finanziarie dell'azienda e che oggi, di fatto, viene riportato alle casse dello Stato. questo è un risparmio del cittadino, e non è più nella disponibilità immediata nel rapporto tra amministrato e amministratore all'interno della società nella quale il lavoratore presta la sua opera perché viene trasportato nelle casse dello Stato, allora si ha, in virtù della trasmigrazione dei fondi, o un prestito (e quindi quel prestito dovrebbe essere onorato, non già per

del convincimento della persona fisica, non lavoratore, ma imprenditore (sappiamo che il reddito delle persone fisiche può benissimo riguardare l'attività di di un cittadino come imprenditore agricolo, come professionista o come società individuale). Infatti, nel momento in cui ho messo a rischio il mio capitale e, coniugando rischio e iniziativa, ho programmato un obiettivo di rendimento di esso, ho certamente considerato, nella prestazione del servizio o nella elaborazione del prodotto di cui alla mia attività, un giusto compenso, per poter far sì che il rendimento del mio capitale sia bastevole anche al pagamento delle imposte.

Pertanto, a questo punto l'accordo a base del rapporto contrattuale di cui alla tassa verrebbe ad avere un perfezionamento riconsiderato al di là della perimetrazione iniziale dell'accordo stesso; ma variando l'accordo, viene ad essere variato il contratto e quindi unilateralmente viene ad essere violentato il perfezionamento che era stato realizzato prima, con l'accordo contrattuale afferente la tassazione. Sono motivi di di evidente contrarietà rispetto alla civiltà giuridica rispetto alla quale, sia nelle discussioni della maggioranza che, evidentemente, nella difesa del cittadino fatta dall'opposizione, ci siamo ritrovati a dover rappresentare i nostri due diversi punti di vista. è evidente che la maggioranza e il relatore addivengono sostanzialmente alla ragione che prospettiamo, di critica alla finanziaria, atteso che l'unica difesa che viene fatta è dal punto di vista procedimentale e non sostanziale. Per questi motivi siamo assolutamente contrari e pregiudizialmente chiediamo un voto di diniego al proseguimento della trattazione del compendio totale, del compendio totale, quindi bilancio e finanziaria, a quest'Aula. Siamo certi che il dibattito che seguirà potrà risolvere alcune delle domande

facendo riferimento alla definizione di politica economica dell'utilizzo di poche risorse, in questa manovra finanziaria ha messo poca volontà, poco intelletto, poco attivismo, poca intelligenza, mentre la volontà degli italiani era per una finanziaria che desse molte risposte, che consentisse molto sviluppo, che bloccasse il declino. Approfitto del fatto che Approfitto del fatto che il Presidente è distratto e ancora non mi toglie la parola per dire, ancora una volta, che la nostra posizione non può essere che contraria, nei modi e nei fatti.

Sono sicuro che ella, Presidente, manterrà salve le prerogative del Senato e non si discosterà dalla prassi che negli ultimi tempi ha visto il Governo porre la questione di fiducia sulle finanziarie su testi precisi, perché attualmente non credo ci sia un testo. A meno che il Governo non voglia porre la fiducia sul testo approvato dalla Camera, infatti, non esiste un testo della finanziaria sul quale fare la questione di fiducia. Il problema del ritardo nell'approvazione e nell'*iter* e nell'*iter* pasticciato di questa finanziaria dipende proprio dalle incertezze, dai ripensamenti, dalle continue revisioni, dal numero imponente di emendamenti che il Governo e la maggioranza hanno portato avanti anche nell'ultima fase dell'esame della finanziaria da parte del Parlamento. In sostanza, ciò che si è verificato in Commissione ha dimostrato con evidenza che il Governo e la maggioranza non hanno la forza parlamentare necessaria per far democraticamente approvare dal Parlamento la legge finanziaria, ma devono far ricorso a un vero e proprio atto di forza per imporre al Parlamento decisioni prese altrove. Si dice che vi sia stato una sorta di ostruzionismo da parte dell'opposizione.

Signor Presidente, normalmente l'esame della finanziaria si conclude in Commissione, anche quando ci sono emendamenti in numero maggiore rispetto a quelli presentati in questa sessione. Ciò non accade, invece, quando da una parte si cerca di conculcare i diritti dell'altra, soprattutto sapendo qual è la reale condizione economica e politico-parlamentare del Paese.

bilancio, del quale chiediamo che sia rinviato e sospeso l'esame: questo bilancio, infatti, è costruito - lo abbiamo visto con chiarezza nell'illustrazione che ieri ha fatto in Commissione il vice ministro Visco - su dati delle entrate che non corrispondono alla realtà dei fatti. Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo perché il Governo si ostini ad impostare una manovra di così ampie dimensioni, tanto che, ad avviso del Governo stesso, essa avrà effetti deflattivi, cioè farà diminuire il potenziale di crescita di reddito nel 2007, in presenza di entrate così cospicue che avrebbero consentito una manovra di minori dimensioni e quindi una maggiore possibilità di crescita del Paese il prossimo anno. L'unica risposta - ahimè, credo, inconfessabile - è che solo una manovra di cospicue dimensioni può consentire al Governo di mascherare, nell'ambito della stessa, una serie di spese e regalie che altrimenti non sarebbero potute essere consentite. Basta vedere gli ultimi 100 articoli del

fantasmagorica somma di oltre 1 miliardo e 600 milioni di spese *à gogo* e non giustificabili; basta vedere le novelle introdotte dalla Camera e gli oltre 150 emendamenti governativi proposti, e poi per fortuna caducati dopo l'esame in Commissione bilancio del Senato, quante e quali regalie contengano. Signor Presidente, delle due l'una: o questo Governo sa di avere i giorni contati e prepara una finanziaria elettorale modello *Ancien régime*, facendo regalie a tutti, a danno dei contribuenti, cosa che non dovrebbe che non dovrebbe essere consentita in questa fase (chiedere più tasse ai contribuenti per finanziarsi una campagna elettorale mi sembra francamente un modo di procedere non condivisibile), oppure non sa più neanche quello che vuole. Infatti, l'episodio

con l'utilizzo dei fondi dormienti, quindi in un modo assolutamente contrario a qualunque regola non solo di contabilità ma di buon senso, significa che l'unico obiettivo della maggioranza è utilizzare la leva fiscale non per risanare il Paese, ma semplicemente per realizzare meccanismi di scambio politico che non sono assolutamente giustificabili in questa fase. È quindi una finanziaria che non serveallo sviluppo, perché troppo cospicua nelle sue dimensioni,

Signor Presidente, questo dibattito offre l'occasione per una riflessione su quanto ha detto in Aula il presidente Morando. Vorrei approfittare di questa occasione innanzitutto per ringraziarlo per il lavoro svolto in Commissione e per come ha assicurato la possibilità a tutti noi di discutere e di svolgere, pur nella confusione generata dalle incertezze e dalle difficoltà della maggioranza, un lavoro il più possibile ordinato. ordinato. Condivido le riflessioni del presidente Morando e sono lieto che egli abbia previsto per la ripresa dei nostri lavori a gennaio una discussione su tutte le regole della nostra sessione di bilancio e sulla formazione della finanziaria sul bilancio dello Stato.

in Parlamento con una finanziaria senza relatore e che sarà quindi approvata con un voto di fiducia su un maxiemendamento. Se non si è arrivati a concludere i lavori in Commissione,

dichiarazioni il ministro Chiti avrebbe sostenuto che non siamo arrivati ad una conclusione perché «l'opposizione aveva fatto ostruzionismo in Commissione bilancio che non ha consentito la conclusione della discussione». Ebbene, in quella dichiarazione del ministro Chiti vi è tutta la malafede del Governo in questa situazione, perché la premessa di tali considerazioni sul ruolo dell'opposizione è che, entro domani, nel pomeriggio, il Governo presenterà il maxiemendamento e chiederà la fiducia. Allora, se la maggioranza era già d'accordo, se dalla cabina di regia era scaturita l'intesa tra i Gruppi ed il Governo, se tutto era pronto, perché il maxiemendamento non è all'attenzione dell'Assemblea già stamattina? Per la semplice, banale ma evidente ragione che la maggioranza ed il Governo non hanno trovato, a partire dal DPEF, fino ad oggi un punto di equilibrio e di accordo al loro interno. Quindi, fino ad oggi abbiamo patito l'ostruzionismo del Governo sulla Commissione e l'ostruzionismo della maggioranza su se stessa. Questa è la verità dei fatti. Se di nuove regole abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di regole che impediscano ai Governi di praticare non soltanto l'ostruzionismo e l'espropriazione del Parlamento, ma anche l'espropriazione della verità rispetto agli italiani. Se infatti si vuol far passare questo voto di fiducia, così come il precedente alla Camera e come il prossimo che ci sarà sempre alla Camera, che il ministro Chiti già dà per scontato, come provocato dall'opposizione, ebbene questa è una menzogna in termini politici ed è menzogna grave che il Governo pagherà con la caduta e il crollo del consenso, che ormai da alcuni mesi si sta verificando. Che la prova del conflitto all'interno della maggioranza sia evidente ce l'ha data oggi con le sue dichiarazioni alla stampa il presidente del Gruppo di Rifondazione Comunista Russo Spena, il quale ha sentito la necessità di dire pubblicamente il Governo deve recepire gli orientamenti della cabina di regia e che nel maxiemendamento siano rigorosamente recepiti gli emendamenti approvati in Commissione bilancio sui primi 17 articoli su quanto è stato discusso dell'articolo 18. Il che lascia presagire con molta chiarezza che il rigore che richiede il presidente Russo Spena al momento manchi assolutamente e che il livello di conflitto in stanze lontane dal Parlamento sia elevatissimo.

possiamo contare sei o sette versioni di leggi finanziarie diverse e ancora non sappiamo - ad oggi - quale sarà la finanziaria definitiva per l'anno 2007.

che è stato, come ho detto prima (grazie anche all'impossibile sforzo, contro la sua stessa maggioranza e il Governo che essa esprime, del presidente Morando), ordinato, approfondito, serio, rigoroso, determinato, ma che - ahimè - si è svolto su un oggetto diverso da quello su cui il Parlamento, il Senato e la Camera nei giorni successivi, voteranno. Se abbiamo un problema di regole, non lo abbiamo tanto sulle modalità di discussione al nostro interno, sul modo con cui queste stanno funzionando

la legge di bilancio, il *budget*, all'approvazione, prendere o lasciare, delle Camere). No: ci siamo arrivati attraverso un costante e ripetuto inganno nei confronti del Paese e delle Camere, secondo il quale dal Parlamento sarebbe dovuto scaturire un testo sul quale, eventualmente, sarebbe stata posta la fiducia. Tutto ciò è stato impedito

da quando è in carica, sta lavorando contro il Paese, contro l'economia e lo sviluppo e che sta ricorrendo ad ogni genere di piccolo ma continuo e ripetuto inganno nei nostri confronti e nei confronti degli elettori, in realtà per dare al Paese una stangata che è frutto della sua ideologia e del coacervo di ideologie che si raggruppano in questa maggioranza, in questo Governo e nella maggioranza politica ed elettorale che lo ha espresso. È in parte un desiderio di vendetta sociale nei confronti di un Paese che vuole cambiare e che ancora oggi non ha lasciato il passo: lo ha dimostrato nelle manifestazioni del 2 dicembre e lo dimostra in tutte le occasioni in cui i Ministri vanno a riscuotere la loro meritata dose di fischi. Il Paese è ormai lontano da questo Governo. Il Governo dovrebbe prendere atto che non è l'opposizione a fare ostruzionismo alla sua azione, ma l'Esecutivo a fare ostruzionismo al Paese. *(Applausi

a parlare il senatore Banti. Come tale, essa impegna politicamente e - vorrei dire - eticamente il nostro Governo a confrontarsi sulle linee di indirizzo che traguardano, anche alla luce della pluriennalità dei documenti di bilancio, l'intera legislatura. Sarebbe dunque sbagliato leggere i documenti al nostro esame (il disegno di legge di bilancio e la legge finanziaria) limitatamente all'anno che abbiamo di fronte, cioè all'esercizio finanziario 2007. invece, leggerli come primo passo di un programma più ampio che traguarda obiettivi importanti di finanza pubblica e di riorganizzazione del nostro Paese.

che l'Aula del Senato, così come l'Aula della Camera dei deputati, ha votato, attraverso la mozione di indirizzo, nello scorso mese di luglio. Il Documento di programmazione economico-finanziaria ha ben chiarito come

e che riguarda specificamente un rapido rientro nel rapporto del 3 per cento tra *deficit* e prodotto interno lordo, come indicatoci dall'Unione Europea, a fronte di un pericoloso e grave sforamento di tale limite

accettati dall'Italia e dal nostro Parlamento ed è nostro dovere, al di là delle difficoltà che di volta in volta si possono manifestare, rientrare in tale perimetro. Ciò però non è sufficiente, dice il Documento di programmazione economico-finanziaria, richiamando il dato macroeconomico del pesante debito pubblico che l'Italia si porta dietro da molti anni: un debito pubblico ampiamente superiore al 100 per cento del PIL e che ovunque ha ripreso a salire negli ultimi due anni. Non si tratta di abbandonarsi in questa sede a polemiche più o meno accese nei confronti di chi ha governato l'Italia negli anni precedenti; resta il fatto che il nuovo Governo, insediatosi alla guida del Paese, si è trovato e si trova di fronte ad una situazione che non è possibile far andare avanti così come si è manifestata nei mesi passati e in corso d'esercizio. Dobbiamo ridurre il debito, che è un pesante macigno sulle nuove generazioni, su tutti noi, sull'economia di questo Paese e sulla possibilità che esso rimanga a testa alta nel novero delle più importanti Nazioni del mondo. È evidente che una riduzione consistente del debito pubblico non può avvenire in corso di un unico esercizio, ma deve traguardare un percorso più lungo, ancorché deciso.

la massa del debito pubblico: la sanità; le pensioni ed il pubblico impiego, gli enti locali. Si tratta di comparti di non poco rilevo nell'ambito dell'organizzazione del nostro Stato; anzi - e

tutto deve essere parametrato all'andamento delle vicende del tempo che ci è dato di vivere e delle prospettive che in esso si aprono, si materializzano e si concretizzano. Gli aggregati della spesa pubblica,

che comprende anche la pluralità degli enti locali e l'insieme del pubblico impiego, sia pure con le sue contraddizioni ed i suoi problemi (come la questione del precariato, che è tuttora all'ordine del giorno, o della funzionalità e della produttività della spesa pubblica, e così via). Tutto ciò richiede azioni di riforma certamente incisive, ma anche concertate - come del resto prevede il programma della nostra coalizione - e, quindi, un tempo adeguato, che si potrà manifestare (come del resto è stato già stabilito, ad esempio, per quanto riguarda il settore delle pensioni) nel corso dell'anno che abbiamo di fronte, il 2007. La legge finanziaria, dunque, ha dovuto procedere alla manovra di rientro sotto il 3 per cento del rapporto *deficit-*PIL senza poter inizialmente prospettare l'insieme degli interventi che devono essere adeguatamente preparati e concertati sui quattro grandi aggregati di spesa. Non credo che questo sia un errore, ma un giusto modo di procedere, che, però, ha portato con sé la conseguenza che gli interventi della legge finanziaria - anche se particolarmente ben congegnati, a mio giudizio - prestano il fianco alle critiche di chi in essi

ed il pubblico impiego, ma non certamente la sanità e le pensioni, settori che richiedono ben più ampi interventi di discussione, anzitutto, e di preparazione nell'ambito delle riforme). riforme). La legge finanziaria e la manovra di bilancio che stiamo discutendo per il 2007, allora, scontano tale necessità di affrontare due tempi e due misure che vanno collegati tra di loro.

di filosofia dello Stato, se così mi posso esprimere, cioè di organizzazione dell'intero Stato italiano. Ciò alla luce di cambiamenti epocali (che sono già avvenuti e che ancora sono in corso), sia per quanto riguarda la globalizzazione del Pianeta (cioè la

degli interventi che devono essere affrontati nell'ambito dei rapporti tra i diversi livelli di presenza della società italiana (a cominciare dal

Oggi siamo in presenza di fenomeni, per certi aspetti, quasi inversi ma di grande complessità che devono essere visti in un'ottica di lungo periodo. Questioni come quella dell'ambiente, quella del rapporto fra centro e periferia,

al governo del Paese, di responsabilità di disastro economico, ma certamente chi ha governato l'Italia nei cinque anni precedenti non può non assumersi la responsabilità di contribuire

potranno aprirsi scenari interessanti dal punto di vista dell'azione complessiva di riordino e di riforma nel nostro Paese, di cui i provvedimenti finanziari attuali costituiscono la premessa.

Dobbiamo evitare che si verifichi quanto avvenne in Italia nel 1876, quando il Governo Minghetti della Destra storica arrivò al pareggio di bilancio imponendo pesanti sacrifici al Paese, ma pochi mesi dopo cadde in Parlamento e venne sostituito dal Governo Depretis. Non c'erano infatti le condizioni perché, a fronte dei sacrifici sostenuti, quella maggioranza e quel Governo continuassero a governare il Paese. non può essere questa. Oggi sappiamo che una maggioranza attenta alle attese popolari può forse dare l'impressione di scontentare qualcuno, ma nella prospettiva di fondo c'è invece l'esigenza

Signor Presidente, colleghe e colleghi del Senato, signori rappresentanti del Governo, mi fa piacere parlare in quest'Aula, insolitamente silenziosa,

per l'economia e per la vita sociale del nostro Paese nel 2007 e anche negli anni successivi. Mi permetto di avanzare alcune considerazioni di carattere generale. Il nostro Paese, sulla scia dell'Europa, ha iniziato una fase di ripresa economica. Sul vigore e sulla durata di questa influiranno alcune riforme sulla cui necessità gli osservatori indipendenti esprimono un giudizio per lo più concorde. Queste riforme non si fanno dalla sera alla mattina ed esigono concertazione e gradualità: alcune sono state predisposte dai primi atti di Governo, altre sono contenute nei provvedimenti che qui discutiamo, altre ancora saranno avviate nel 2007. Riforme che debbono mirare ad aumentare l'efficienza del Paese, ad innovare e ad accrescere il patrimonio di conoscenze, a rafforzare le infrastrutture, a ridurre in modo permanente ed irreversibile l'evasione fiscale, a far emergere le attività al nero, a far crescere le persone attive (perciò creatrici di reddito e ricchezza) in rapporto alla popolazione. Riforme, insomma, che facciano salire di qualche gradino la funzionalità del Paese: ci si può certo dividere sui metodi da seguire per avviarle e realizzarle, ma pochi, credo, dissentono sulla loro utilità e sulla loro finalità. Che posto ha il sistema di *welfare* nell'efficienza e nella crescita di un Paese? Molti ritengono che esso appesantisca lo sviluppo, attenui la competitività, scoraggi l'iniziativa, trasferisca troppe risorse da chi produce ricchezza a chi è incapace di farlo. Sotto questo profilo, il sistema europeo è messo sotto accusa, poiché si collega il lento sviluppo dell'ultimo decennio con quello più dinamico degli Stati Uniti, dove lo Stato sociale è assai meno generoso. Tuttavia, questa diagnosi è superficiale e non tiene conto che nell'arco dell'ultimo mezzo secolo la *performance* europea è stata migliore di quella americana e che un continente piccolo e densamente popolato come l'Europa, con fitti rapporti sociali, variegati e levigati da una storia di millenni, con una lunga storia di miseria, povertà e disuguaglianza, esprime una forte domanda di tutela sociale che, invece, il giovane, vasto, aperto e ricco continente americano può, in certa misura, ignorare. La storia, dunque, consiglia avvedutezza nella riforma dei sistemi sociali; non è scritto in nessun sacro testo che il Paese che trasferisce ics più uno per cento al sistema di protezione sociale debba avere uno sviluppo frenato rispetto a quello che trasferisce solo l'ics Non è scritto in alcun sacro testo che una distribuzione del reddito e della ricchezza meno egualitaria - come avviene in America - sia più favorevole allo sviluppo di quanto lo sia una distribuzione meno disuguale, tipica dell'Europa. Nella competizione della crescita l'Europa può continuare ad essere Europa, e l'America America, e giocarsi su altri fronti la partita. L'Italia, come è noto, trasferisce una quota di PIL con finalità di protezione sociale che è, più o meno, in linea con quella dei maggiori Paesi dell'Europa continentale. Tuttavia, è opinione comune che vi sia una distribuzione inefficiente, e per certi aspetti iniqua, dei trasferimenti sociali, e questa finanziaria, cui non compete il compito di riformare il sistema, va giudicata valutando se i suoi meccanismi attenuino distorsioni e disuguaglianze e se facilitino il cammino delle necessarie riforme. Mi soffermerò su tre punti significativi, seppure di diversa portata economica. Si consideri la revisione delle aliquote IRPEF, l'aumento delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia e la rivalutazione degli assegni per il nucleo familiare. Nell'insieme, queste misure operano un consistente trasferimento di risorse alle famiglie con figli, valutabile attorno ai 3 miliardi di euro, con una redistribuzione, sia pure moderata, a favore delle famiglie meno abbienti. Nell'insieme è una benvenuta inversione di tendenza, se si pensa che il secondo modulo della riforma fiscale del Governo Berlusconi aveva avuto un effetto redistributivo regressivo: nella struttura universitaria della quale ero parte, la riforma IRPEF aveva restituito al sottoscritto, all'apice della carriera, una somma equivalente ad oltre dieci volte quanto era stato restituito al dipendente di grado più basso, nonostante il mio stipendio fosse di quattro volte più elevato. L'aumento degli assegni per il nucleo familiare è un altro segnale benvenuto: ricordo che, tra i Paesi dell'Unione Europea, l'Italia è quello che trasferisce meno risorse pubbliche, in termini sia assoluti che relativi, al settore denominato «famiglie e figli»: per cento della spesa sociale, contro il 5-6 per cento nella media e il 10-12 per cento della Francia e dei Paesi scandinavi. Ci attendiamo però che, dopo la finanziaria, si cominci a metter mano ad un programma di legislatura per la riforma del sostegno alle famiglie, dal quale sono cospicuamente escluse le famiglie incapienti, almeno un milione, e quelle che non hanno titolo a ricevere l'assegno per il nucleo familiare perché autonomi o precari. La riforma dovrà tendere a realizzare un sistema di integrazione del reddito alle famiglie con figli e con redditi medio-bassi di tipo universalistico, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. Esiste, a questo proposito, un menù un menù di valide proposte cui il legislatore può attingere. Una riforma che dovrebbe anche includere, secondo quanto stipulato dal programma dell'Unione, una misura universalistica a favore di ogni nato volta a dotarlo, alla maggiore età, di risorse che ne favoriscano l'indipendenza, l'autonomia e una più veloce transizione all'età adulta. Il secondo significativo segnale che mi preme sottolineare riguarda il piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, con l'obiettivo di raggiungere nel 2010 una copertura quadrupla dell'attuale, e pari al 33 per cento, dell'universo infantile sotto i tre anni. Lo stanziamento di 100 milioni annui, per il triennio 2007-2009, andrà ripartito fra le Regioni in sede di Conferenza unificata. Segnalo questo intervento - ma altri ve ne sono non meno rilevanti, quali il finanziamento del fondo per le politiche della famiglia e quello per le pari opportunità - perché affronta, in modo finalmente concreto, il tema della sottodotazione di strutture e servizi per l'infanzia e che vanno, in definitiva, a beneficio delle famiglie. Vale la pena ricordare, tra l'altro, che la natalità del Paese rimane bassissima, nonostante il contributo crescente della popolazione immigrata. Sostenere la natalità, oggi, significa non solo fornire integrazioni di reddito per chi ha responsabilità genitoriali, ma anche erogare più servizi per i bambini, favorire un'equilibrata ripartizione di oneri e funzioni tra i generi, assicurare davvero alla donna che ha figli da allevare uguali opportunità di lavoro e di carriera, rispetto a chi non ha queste responsabilità o ne ha in misura minore. Nella società del 2000, il fatto che la donna percepisca un reddito autonomo e stabile è garanzia di decisioni riproduttive serene ed equilibrate, mentre la mancanza o l'incertezza di reddito proprio è causa di rinvii o rinunce. Questi positivi segnali di attenzione verso genitori e figli vanno sicuramente rafforzati, integrati e coordinati, evitando di scivolare sulle bucce di banana della definizione di «famiglia». Ogni bambino ha diritto ad un equo sostegno, indipendentemente dalla condizione, origine, genere di chi ha responsabilità genitoriali. Quanto al terzo e ultimo punto, l'immigrazione è la maggior fonte di cambiamento sociale in questi primi decenni del secolo. Il 6 per cento della popolazione del Paese è immigrata e contribuisce al 7 per cento del PIL nazionale; immigrato è il 10 per cento dei lavoratori ed i figli con almeno un genitore straniero sono il 12 per cento Queste proporzioni sono in rapida crescita. Un fenomeno di questa portata deve essere governato, senza risparmio di risorse, nel suo aspetto più delicato: quello dell'integrazione. La creazione di un fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, alimentato da 50 milioni annui nel triennio 2007-2009, è un modesto segnale di salutare inversione di marcia, rispetto al precedente Governo che non aveva rifinanziato il fondo per l'integrazione previsto dall'articolo 45 del testo unico sull'immigrazione. La materia andrà ripresa con vigore in sede di revisione della legislazione sull'immigrazione e di gestione delle politiche migratorie: segnalo solamente che 50 milioni sono assai pochi e si commisurano a meno di 200 euro per ogni nuovo immigrato, o a meno di 20 euro per componente dell'intero *stock* di immigrati. Le risorse necessarie per sostenere le politiche di accoglienza, inserimento, inclusione, integrazione e interazione tra immigrati, i loro figli e la società ospitante sono sicuramente molte di più. Ho voluto sottolineare questi tre aspetti non tanto e non solo per le risorse messe in campo, ma perché segnalano la volontà di muoversi nella giusta direzione. Un solido sviluppo non viene assicurato da meno *welfare*, ma da un *welfare* più efficiente e più giusto. È anche per questo che, in consonanza con il Gruppo cui appartengo, darò voto favorevole alle leggi che andremo a votare. *(Applausi dal

La diversità sta nella condizione per cui stiamo discutendo sul bilancio, di fatto anticipando una parte della discussione che

ne fanno risaltare le contraddizioni, sollecitando la dialettica, la ricerca della permanenza nel vario e l'accordo tra le diverse opinioni, il numero di emendamenti denota che sul bilancio non c'è questa necessità: si tratta di cinque emendamenti al bilancio. E allora perché stiamo parlando di bilancio? *In primis*, perché il bilancio, in una discussione che già da qualche tempo (per noi, in quella speciale accademia che è la Commissione bilancio, per gli altri forse con considerazioni di una certa sterilità),

che la nostra intenzione è quella di modificare la legge di bilancio, in quanto non è possibile che in essa si effettuino richiami sostanziali. Se si fanno nella legge di bilancio, legge formale, richiami sostanziali significa che questa ha fallito il suo obiettivo.

devono essere coinvolgenti il Parlamento ed attivate dalla conoscenza che il Parlamento deve avere sull'attività del Governo, dice: quello che si fa a seguito di questa disposizione deve essere messo a conoscenza del Parlamento attraverso le Commissioni permanenti.

una valutazione di merito, quanto inserito e disposto nella legge di bilancio non dovrebbe essere sottoposto, in quanto disposto dalla legge di bilancio, alla valutazione di merito delle Commissioni Quindi questo bilancio, ma non soltanto questo, acuisce, esalta, porta al suo termine una patologia sempre più febbrile della strutturazione della legge di bilancio. La legge di bilancio e la legge di contabilità non hanno avuto un tradimento sostanziale.

e questo dibattito si è aperto nel Paese - in una democrazia che, indipendentemente da ciò che si vuole, nella sua materialità è novellata, molto ma molto fortemente, in modo presidenziale. Mentre la democrazia è novellata in senso presidenziale, le norme di contabilità sono proprie di una democrazia parlamentare. Quindi il Governo, che prima trovava giustificazione nella questione di fiducia soltanto in certi momenti, oggi ha una deriva per cui finisce per avere una giustificazione politica a porre la fiducia sempre e più costantemente.

deriva dalle necessità attuale ed è giustificata dalle prerogative che la novella della Costituzione in senso presidenzialista ha dato per cui un Governo forte - perché ha un mandato popolare,

non me ne vogliano i colleghi della maggioranza - e di fatto non ritiene fortemente importante che essa sia esitata da un voto della Commissione: se così fosse, ad esempio, nella fase in cui siamo riusciti a

nelle famose sette questioni di fiducia poste con le manovre finanziarie del 1992) emanata dalla Presidenza del Consiglio, di cui Amato era sottosegretario, che diceva che la legge, quando vi è un articolo, deve avere una serie di disposizioni coerenti ed omogenee per finalità. In questo senso abbiamo emanato questi 17 articoli ed abbiamo avuto, però, la netta sensazione che il Governo non fosse estremamente attento a valutare nel senso che declinava nei confronti degli emendamenti della maggioranza una valutazione favorevole e quindi a questo punto una loro approvazione ed un ricevimento nella legge finanziaria. Perché questo? In definitiva è evidente che non vi era nessun motivo di aprire le maglie

a una riforma della legge di contabilità una delle cose possibili e doverosamente fattibili da parte nostra è obbligare ad un esito definitivo (se non in Aula, perché deve essere salvaguardata la prerogativa del Governo di avere la fiducia dalla propria maggioranza), cioè alla necessità che tutta la finanziaria venga discussa in in Commissione. Non è soltanto un motivo di discussione speciosa del quale finiamo per parlare perché ci dilettiamo di questi problemi. È evidente che uno dei uno dei sali della democrazia è il fatto che se io opposizione mi confronto con la maggioranza, dal numero, dalla quantità e dalla più o meno pervicace intenzione della maggioranza di difendere o no una norma posso capire e percepire la sensibilità della stessa rispetto ad un problema e quindi misurare la mia capacità di intervento rispetto alle iniziative da predisporre a favore dei cittadini (lo stesso per quanto riguarda la maggioranza). Quindi, Quindi, ci richiamiamo ad una necessità che se non viene salvaguardata, se non viene riaffermata, finisce per recare nocumento al procedimento di formazione della legislazione finanziaria e quindi alla politica economica. Quella politica economica sarebbe infatti determinata da un compendio legislativo

obbligatoriamente la definizione e il perfezionamento della parte formativa, pregiudiziale all'esito definitivo. Quindi, deve esserci una sostanziale e pedissequa analisi, senza la quale verrebbero ad essere tradite le intenzioni che che nella stesura della legge di contabilità erano intestate all'altro sistema e che erano assoluta garanzia di trasparenza, almeno nelle intenzioni. Quindi un perfezionamento del procedimento che fosse quanto più rispondente alle intenzioni del legislatore nell'interesse del cittadino.

un documento firmato da 52 senatori con cui chiedevamo la riduzione delle spese per gli armamenti e, contemporaneamente, la creazione di un fondo per la riconversione produttiva al civile.

(sono stati tolti 50 milioni su 3.257: è un dato che apprezziamo, anche se non lo riteniamo sufficiente).

PIL alla spesa sociale, in Germania l'8,3, senza contare che di parte della spesa sociale - com'è giusto, ovviamente - godono gli stesso familiari dei militari: servizi per l'infanzia, l'istruzione e i trasporti pubblici. Per non citare le spese molto inferiori in Italia per l'università e la ricerca. Ci saremmo aspettati almeno che questa finanziaria mettesse in discussione, all'interno del capitolo della difesa, la suddivisione fatta tra le spese per gli armamenti e le spese per l'esercizio. Di fronte a una spesa per l'esercizio decisamente inferiore alle necessità quotidiane e alle reali esigenze delle nostre Forze armate, che significa difficoltà ad affrontare manutenzione e addestramento

al 21,8 del 2007. Dunque, il Governo del centro-sinistra ha quasi raddoppiato le spese per gli armamenti. Questo aumento così vistoso è politicamente inaccettabile, soprattutto in coerenza con il programma dell'Unione che prevede una «riduzione degli armamenti»: questo patto dovrebbe legare tutta la maggioranza. In Commissione difesa, dove ho sollevato il problema, mi è stata risposto: sono impegni già presi dal Governo precedente che noi dobbiamo onorare. Questo non giustifica però la trasgressione del nostro patto: può essere politicamente più conveniente pagare penali, uscire dai contratti o ridurne la portata, piuttosto che dover affrontare nei prossimi anni ulteriori e maggiori spese per armamenti non indispensabili.